L'azienda si trova ad affrontare una situazione connotata dalla difficoltà di mantenere le proprie quote di mercato in ragione del notevole abbassamento del prezzo del prodotto venduto. Del resto, il consumo di nylon, prodotto principale della società, è in costante diminuzione rispetto al consumo mondiale di fibre (a fronte di un aumento del consumo mondiale del poliestere, della lana e del cotone). Quanto descritto influisce sullo sfruttamento degli impianti di produzione del nylon a livello mondiale, il cui utilizzo si attesta su una percentuale prossima al 60 per cento rispetto all'80 per cento degli scorsi periodi. In tale contesto generale, la Radici Yarn ha visto diminuire la propria quota di mercato nel corso degli ultimi due anni, il che ha conseguentemente portato ad una sottoutilizzazione degli impianti. La società ha, pertanto, chiesto ed ottenuto la concessione, per un periodo di 12 mesi decorrenti da marzo 2009, di un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria, per fronteggiare un periodo di forti difficoltà dovuto principalmente al pesante calo degli ordinativi. In particolare, lo stabilimento di Pistoia è interessato totalmente dalla cassa integrazione guadagni in quanto legato ad un settore di monoproduzione, ovvero filo nylon per calza, diversamente dallo stabilimento di Villa d'Ogna in che ha subito una riduzione parziale della produzione, essendo la stessa diversificata per differenti tipologie di prodotti. Si informa, altresì, che è in atto una riconversione di alcune linee produttive dello stabilimento di Villa per far fronte alle residue richieste del prodotto precedentemente realizzato nello stabilimento di Pistoia. Per quanto riguarda, appunto, lo stabilimento di Pistoia, la Regione Toscana ha convocato le parti, a fronte della volontà della società in questione di cessare l'attività del sito produttivo, con l'obiettivo del raggiungimento di un accordo per la corresponsione di incentivi a favore dei lavoratori e per individuare forme di deindustrializzazione del sito produttivo. L'esame si è articolato in due successivi incontri, il 17 giugno 2009 e il 23 giugno 2009, con la presenza dell'azienda, dei rappresentanti dei lavoratori e delle istituzioni (oltre alla Regione erano presenti la Provincia di Pistoia ed il Comune Dopo una complessa ed articolata trattativa, tuttavia, si è dovuto prendere atto che le posizioni rimanevano distanti; in esito al mancato accordo, la società ha avviato la procedura di mobilità per l'intera forza lavoro. Il Ministero dello sviluppo economico ha comunicato la disponibilità a convocare le parti interessate, al fine di discutere di un possibile protocollo di intesa che contempli misure volte a facilitare progetti di reindustrializzazione. vorrei rassicurare gli interroganti in ordine all'attenzione con la quale il Governo segue la vicenda con l'impegno a fornire notizie in ordine agli ulteriori sviluppi della situazione descritta.

vengono riconvertite nell'altro stabilimento. Comunque, il problema, non è questo, anche se vi sono delle contraddizioni: ci sono stati in questo stabilimento investimenti da parte della proprietà per circa 8 milioni di euro, realizzati non 15 anni fa, ma tra il 2007 e la fine del 2008; cioè, fino ad un anno fa si è investito dai 6 agli 8 milioni di euro. In

In quegli incontri, infatti, sono stati definiti ammortizzatori sociali e strumenti risarcitori che potranno durare due anni. Questo è il punto che sottopongo alla sua attenzione, signor Sottosegretario:

Presidente, va in premessa detto, nel rispondere a questa interrogazione, che il terminale *offshore* per la ricezione, lo stoccaggio e la rigassifìcazione del gas naturale liquefatto

relativa alla prevenzione ed alla riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) ed è pertanto soggetto ad autorizzazione integrata ambientale (la cosiddetta AIA), di competenza statale, ai sensi dell'allegato V, punto 6), del decreto legislativo n. del 2005, in quanto si tratta di impianto localizzato interamente in mare. Sulla base di quanto dichiarato dal gestore in sede di domanda di AIA, sul terminale risulta svolta l'attività prevista al punto 1.1, quella cioè di impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 megawatt, dell'allegato I al decreto legislativo n. 59 del 2005. L'avvio del procedimento è stato comunicato al gestore con nota del 17 dicembre 2007. L'istruttoria tecnica, che ha preso in considerazione anche le altre attività connesse condotte sulla piattaforma, è stata svolta dalla commissione istruttoria per l'autorizzazione integrata ambientale - IPPC. Sulla base del parere tecnico conclusivo reso dalla commissione in data 10 dicembre 2008, si è tenuta presso il Ministero dell'ambiente la seduta della Conferenza dei servizi, convocata ai sensi dell'articolo 5, comma 10, del decreto legislativo n. 59 citato, che si è espressa favorevolmente in merito al rilascio dell'AIA, ma con prescrizioni. Pertanto, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in data 21 gennaio 2009, è stata rilasciata l'autorizzazione integrata ambientale di durata quinquennale dalla data del rilascio. Copia del provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni è messa a disposizione del pubblico per la consultazione, nell'apposito portale *web* della Direzione salvaguardia ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,

recante attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo degli incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (si tratta della cosiddetta direttiva Seveso). L'istruttoria tecnica per la valutazione del rapporto definitivo di sicurezza, di competenza del comitato tecnico regionale del Veneto, risulta conclusa positivamente in data 28 novembre 2008. Ai sensi dell'articolo 7, comma 8, del citato decreto legislativo n. 59 del 2005, le prescrizioni contenute nel parere tecnico conclusivo costituiscono quindi parte integrante dell'AIA. Riguardo alle prescrizioni formulate dalla Capitaneria di porto di Chioggia con propria ordinanza di polizia marittima, si rappresenta che l'interdizione dell'area circostante la piattaforma persegue finalità relative alla sicurezza della navigazione ed alla salvaguardia della vita umana in mare ed ha, per effetto, il solo scopo di prevenire possibili incidenti, definendo un'area operativa di manovra riservata alle sole gasiere ed ai mezzi di servizi tecnico-nautici di rimorchio ed ormeggio, instradando, pertanto, al di fuori di essa le ordinarie rotte utilizzate dalle unità mercantili dirette e/o provenienti dai porti dell'Alto Adriatico e le restanti attività marittime, sia a carattere ludico che professionale (diporto o pesca). Entrando nel merito dei provvedimenti adottati dalla Capitaneria di Chioggia con le ordinanze n. 63 e n. 64 del 2008, si precisa che la predetta area non è pari a 5 chilometri di raggio, ma, come chiaramente evidenziato nella premessa dell'ordinanza n. 64 del 2008, si compone, in dettaglio, di due aree di interdizione concentriche: la maggiore, corrispondente ad una circonferenza di 1,5 miglia nautiche di raggio, è centrata sul terminale GNL; una seconda, più ridotta, di raggio pari a 2000 metri, è anch'essa centrata sul terminale. Nello specifico, si sottolinea che i suddetti limiti dimensionali trovano fondamento nella circolare dell'IMO (International Maritime Organization) n.1/Circ. 257 dell'11 dicembre 2006, recante "Misure di regolamentazione del traffico in aggiunta agli schemi di separazione". L'annesso a detta circolare definisce, infatti, nel dettaglio, l'ubicazione e le dimensioni delle aree di interdizione circostanti ad infrastrutture analoghe a quella in esame, al fine di garantire la sicurezza delle unità in transito nella zona di mare. Da ultimo, si rappresenta che l'ARPA Veneto ha fatto presente che verranno messi a disposizione tutti i dati delle rilevazioni ambientali effettuate dalla stessa Agenzia nell'ambito delle attività di monitoraggio ambientale effettuate, sia a titolo di attività istituzionale che di attività specifica conseguente alla realizzazione del terminale di cui trattasi.

le rilevazioni che si fanno in via teorica e un conto sono, invece, gli effetti che si dispiegano a seguito dell'entrata in funzione di un impianto così complesso. Lo dico con grande tranquillità, anche perché il piano di predisposizione dei rigassificatori è stato approntato dai Governi di centrosinistra e dai Ministri di quello schieramento: quindi, non vi è una contrarietà pregiudiziale. Vi è però l'esigenza, siccome questo è il primo

infatti delle aree marine molto pregiate; vi sono problemi di ripopolazione della fauna ittica;

La messa in funzione e l'inizio degli effetti dell'impianto di rigassificazione e della produzione di questo bene energetico hanno bisogno, proprio per l'unicità dell'impianto, di avere a disposizione delle strutture uniche di accompagnamento e di e di monitoraggio. Lo dico anche perché questo può servire a rassicurare le popolazioni che dovranno ospitare gli altri rigassificatori che sono nel programma di completamento della rete dei rigassificatori nel nostro Paese; diversamente

In ogni caso, un danno economico è stato prodotto; le categorie economiche lo hanno più volte fatto presente al Governo. C'è bisogno di sapere come si accompagna il riposizionamento del sistema economico delle imprese sia di pesca che di turismo: siamo

avente titolo alla stabilizzazione tenendo conto dei principi e dei contenuti degli esiti della verifica ispettiva effettuata dal Ministero della funzione pubblica tra luglio e agosto 2008. Con l'articolo 3 del decreto-legge del 30 dicembre 2008, 208, intitolato «Funzionalità dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale», è stato stabilito: «L'articolo 1, comma 347, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, 24 dicembre 2007, n. 244, si interpreta nel senso che l'autorizzazione ad assumere ivi prevista spiega effetto nei confronti dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) fino al completamento delle relative procedure, a condizione che le stesse siano concluse entro il 31 dicembre 2009». Sulla base di tale novella normativa e in conseguenza degli esiti di una nuova ispezione dei competenti uffici del Ministero della funzione pubblica, azione necessariamente avviata per verificare la regolare attribuzione anche al personale ex ICRAM dello *status* di stabilizzando, con disposizione commissariale n. 382

di conversione del decreto-legge del 30 dicembre 2008, n. 208, l'ISPRA ha previsto l'assunzione, a far data dal 1° giugno 2009, di 201 unità di personale, già a tempo determinato, avente i requisiti di legge per la stabilizzazione. Sulla base di tali azioni e atti amministrativi concreti si è dimostrato, definitivamente, di aver tenuto in massima considerazione gli esiti della procedura selettiva avviata dall'ex APAT con concorso pubblico nazionale, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale, n. 89 del 9 novembre 2004, con l'assunzione a tempo indeterminato del personale altamente qualificato vincitore di quel concorso all'epoca bandito per posizioni di lavoro a tempo determinato. L'ISPRA, dunque, in esecuzione delle disposizioni normative introdotte dalla legge finanziaria 2007 e dalla legge finanziaria 2008 in materia di stabilizzazione del personale precario, ha proceduto all'assunzione di tutto il personale che, in base alle predette disposizioni, era qualificato come stabilizzabile, in quanto in possesso dei requisiti richiesti dalla vigente normativa. proposito, vanno annoverate le disposizioni n. 399 del 10 dicembre 2007 e n. 382 del 30 aprile 2009, con le quali è stata disposta l'assunzione, a far data rispettivamente dal 18 dicembre 2007 e dal 1° giugno 2009, di complessive 325 unità di personale. L'ulteriore personale che permane in servizio con contratti flessibili, ai quali non è possibile applicare le norme sopra citate in materia di stabilizzazione, per carenza dei requisiti richiesti, trova la sua copertura o in progetti finanziati con risorse esterne al bilancio, o in contratti a tempo determinato stipulati ai sensi della normativa recata dal decreto legislativo n. 368 del 2001.

con cui si stabilisce: «Per fare fronte ai propri compiti istituzionali ed alle esigenze connesse con la protezione civile, fino al 30 giugno 2009 l'ISPRA è autorizzato, con oneri a carico del relativo bilancio, ad avvalersi del personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto con contratto di collaborazione coordinata e continuativa». Considerata la scadenza del termine ivi previsto, e cioè il 30 giugno 2009, da quella data il suddetto personale ha cessato il suo rapporto di collaborazione con questo Istituto.

che però mi lascia totalmente insoddisfatto. L'elencazione di una serie di riferimenti, che dal punto ragionieristico e formalistico hanno la loro precisione e fondatezza, non può cancellare il fatto che molte centinaia di lavoratori dell'ISPRA vivono sulla loro pelle e che è davanti agli occhi di tutti coloro che seguono le vicende della ricerca pubblica in Italia: dal 30 giugno di quest'anno, 200 lavoratori precari dell'ISPRA sono stati estromessi dal lavoro e altrettanti ne verranno estromessi entro la fine di quest'anno. Stiamo parlando di una quantità quantità e qualità di risorse umane che, anche in termini percentuali, ha un peso molto significativo sull'ISPRA, sulle sue funzioni, sull'efficacia del ruolo che quell'Istituto L'estromissione di questi 200 lavoratori dopo il 30 giugno è avvenuta, tra l'altro, in un clima molto pesante. Dal giorno dopo, dal 1° luglio 2009, a persone che da anni frequentavano l'ISPRA è stato impedito fisicamente, sulla base di circolari interne del commissario, di raggiungere quelli che fino al giorno prima erano i loro computer, le loro scrivanie.

a tenere alto il nome della ricerca pubblica e dei controlli ambientali nel nostro Paese. Credo che, se non altro dal punto di vista umano, avrebbero meritato e meriterebbero ben altro trattamento. A questo punto, occorre capire se il Ministro e il Governo intendono onorare i loro impegni. Il ministro dell'ambiente Stefania Prestigiacomo, in più occasioni, ha assicurato ai sindacati e ai lavoratori precari dell'ISPRA che, in particolare utilizzando la possibilità di confermare i contratti in scadenza su progetti a valere su risorse esterne,

il comportamento che il Ministro dell'ambiente e il Governo nel suo complesso hanno tenuto e stanno tenendo nei confronti di un pezzo significativo delle tecnostrutture pubbliche italiane sia davvero vergognoso e scandaloso, per motivi sostanziali che riguardano l'importanza di questo settore della ricerca e dei servizi d'interesse pubblico. L'APAT, che oggi è diventata ISPRA, svolge funzioni decisive nell'interesse dei cittadini, per la difesa della loro salute e per la verifica dei livelli di inquinamento; essa inoltre coordina l'attività delle agenzie ambientali regionali. Questo sistema, che è nato alcuni anni fa, ha tanti problemi e tante difficoltà, ma rappresenta una risorsa straordinaria per il nostro Paese. Il Governo Berlusconi, dall'inizio del suo cammino, si direbbe quasi che si sia impegnato sistematicamente per penalizzare questa parte così importante della pubblica amministrazione del nostro Paese. Dietro le chiacchiere e gli annunci del ministro Brunetta sulla necessità di punire i fannulloni, in realtà, si è nascosto un intervento quasi sistematico per impoverire i centri della ricerca pubblica e i centri

Menia, pregando di trasmetterlo anche al ministro Prestigiacomo - che le promesse che sono state fatte, in questo caso ai lavoratori dell'ISPRA, in altri casi ai lavoratori di altre strutture di ricerca pubblica, vengano onorate

vicende. L'indagine denominata "Black mountains", condotta dalla procura di Crotone, con il supporto operativo del Nucleo investigativo sanità e ambiente e della squadra mobile della Polizia di Stato di Crotone, ha portato, il 25 settembre 2008, al sequestro preventivo, su ordine emesso in data 22 settembre 2008 dal Gip del tribunale di Crotone, di 18 aree ubicate nei Comuni di Crotone, Cutro (Kr) e Isola Capo Rizzuto dove gli indagati, dal 1999 ad oggi, avrebbero realizzato vaste discariche non autorizzate di rifiuti pericolosi (circa 350.000 tonnellate), effettuando lavori con l'impiego di materiali tossici costituiti da CIC (conglomerato idraulico catalizzato) e da "scoria cubilot", un composto di sabbia silicea, loppa di altoforno e catalizzatori, (il cubilot) altro non è che un rifiuto proveniente dalla lavorazione delle ferriti di zinco, effettuata nello stabilimento della ex società "Pertusola sud" di Crotone, oggi "Syndial Nel corso dell'indagine, che si ricollega ad un procedimento penale risalente al 1999, condotta dal sostituto procuratore Bruni della procura della Repubblica di Crotone, si è proceduto a nuovi carotaggi sui siti già oggetto di accertamenti. A tutti gli indagati, a seguito delle ulteriori analisi effettuate sui siti indicati, è stato contestato di aver concorso, o comunque cooperato, alla realizzazione di vaste discariche non autorizzate di rifiuti pericolosi

Tra le aree oggetto del provvedimento di sequestro sono ricompresi suoli su cui sono stati costruiti due edifici scolastici, un'area nei pressi della questura di Crotone e la banchina di riva del porto commerciale. inoltre che, in data 17 gennaio 2009, il Gip del tribunale di Crotone ha disposto il sequestro preventivo del suolo e del sottosuolo relativo alle particelle catastali interessate dal tracciato di via Leonardo da Vinci, ad esclusione della strada asfaltata. Tale sequestro è stato disposto sulla base di analisi di campioni, prelevati dalla polizia giudiziaria, ed effettuate dall'ARPACAL di Catanzaro, che accertava che i materiali sospetti rinvenuti avevano una composizione compatibile con "ferriti di zinco" (codice CER 11.02.02: rifiuti della lavorazione idrometallurgica dello zinco classificati come rifiuti pericolosi) "scoria cubilot" (codice CER 10 10 03) e "rifiuti prodotti" da reazioni a base di calcio. Si accertava, dunque, che la ex strada consortile conteneva e contiene, sotto lo strato di bitume, una notevole quantità di rifiuti speciali pericolosi bioaccumulabili (contaminati da zinco, cadmio, manganese, arsenico, piombo, fosforo, vanadio), abbancati senza autorizzazione ed in totale spregio di ogni norma cautelare volta ad evitare la loro diffusione nell'ambiente circostante. Inoltre, in data 11 maggio la predetta autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo del soprasuolo e del sottosuolo relativo ad altre cinque nuove aree ubicate nel Comune di Crotone, per gli stessi motivi di cui sopra. Il fascicolo processuale, atteso che le attività sono ancora nella fase delle indagini preliminari, è secretato e, pertanto, non è possibile fornire ulteriori notizie in merito. Occorre, al riguardo, rammentare che la situazione ambientale della Regione Calabria è critica da almeno un decennio: nel 1997 fu già dichiarato lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani con apposito decreto Da allora si sono succedute varie ordinanze) con le quali sono stati attribuiti ai diversi commissari (ne sono stati nominati già otto) i necessari poteri straordinari, volti a garantire gli interventi dovuti per smaltire detti rifiuti speciali e pericolosi, per approntare la bonifica ed il risanamento ambientale dei suoli e dei sedimenti inquinati, dei siti industriali e delle falde, nonché le operazioni a tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione. Lo stato di emergenza nei termini citati sarebbe cessato il 31 ottobre 2007; poi, con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3645 del 22 gennaio 2008, è stato affidato al prefetto Montanaro il compito di provvedere fino al 30 giugno 2008, in regime ordinario ed in termini di urgenza, al completamento di tutte le iniziative ancora di propria competenza, già programmate ed in corso di attuazione per il definitivo superamento del contesto di criticità ambientale della Regione. Con ordinanza n. 3690 del 4 luglio 2008, l'incarico di Commissario delegato è stato infine affidato al prefetto Goffredo Sottile fino al 31 dicembre 2008 e fino a quella data il Commissario delegato ha costituito a tutti gli effetti il centro di imputazione di diritti ed obblighi. ministri del 18 dicembre 2008 è stato prorogato fino alla fine del corrente anno lo stato di emergenza nella Regione Calabria unicamente nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani.

Con riferimento alle scorie cubilot, in particolare, la procura della Repubblica presso il tribunale di Crotone già il 17 marzo 2004 notificò «la presenza di siti inquinati ai sensi dell'articolo 8 del decreto ministeriale allegando «l'elenco dei siti interessati all'interramento delle scorie di lavorazione del reparto cubilot della Pertusola di Crotone». Ad oggi, dunque, in base alle indagini, risulta la presenza di tale materiale in massiccia quantità, utilizzato per la realizzazione di rilevati e sottofondi stradali, come già indicato, per la costruzione della banchina di riva del porto commerciale di Crotone, presso la discarica di località Armeria di Crotone e, addirittura, risulta impiegato perfino nei complessi contenenti due istituti scolastici. La situazione, pur grave e delicata, è tenuta sotto controllo da parte del Ministero dell'ambiente che, così come in passato, sta tuttora espletando l'attività istruttoria nell'ambito delle Conferenze di servizi relative al SIN di Crotone. In tali sedi è stato richiesto, tra l'altro, all'ufficio del Commissario di accelerare gli studi del gruppo di lavoro per l'indagine epidemiologica da svolgersi sulla popolazione, presumibilmente influenzata dalle attività industriali condotte nel territorio dei Comuni di Crotone, Cassano allo Ionio e Cerchiara Calabra. Non solo. Per il recupero del danno ambientale cagionato, nel 2006 il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, unitamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Commissario delegato per l'emergenza ambientale, ha promosso innanzi al tribunale civile di Milano azione risarcitoria per i danni provocati dall'attività industriale svolta dalla "Pertusola Sud Spa" (oggi "Syndial Spa") nel Comune di Crotone ed in quelli limitrofi. Nell'atto di citazione con il quale è stata introdotta la causa è fatto espresso riferimento alla presenza, fra i contaminanti individuati nell'area Pertusola, di arsenico contenuto, fra l'altro, nelle scorie cubilot. Nel corso dell'istruttoria del procedimento civile, il giudice, con ordinanza del gennaio 2008, ha disposto una perizia tecnica d'ufficio per l'accertamento definitivo dei danni arrecati. Intanto, con ordinanza n. 196 del 25 settembre 2008, il sindaco del Comune di Crotone ha ordinato ai soggetti indagati, nell'ambito dell'indagine sopra citata, di presentare un progetto complessivo per addivenire alla completa bonifica delle aree interessate dal sequestro giudiziario. del territorio e del mare si è immediatamente attivato secondo un principio di precauzione per verificare all'interno dell'area SIN gli interventi di messa in sicurezza da effettuare eventualmente sui siti inquinati, operando in raccordo con il commissario delegato. Anche la causa civile sta proseguendo con la produzione, da parte del Ministero, di ogni elemento ulteriore acquisito. Pertanto, il Ministero dell'ambiente, attraverso la Direzione competente, sta operando per accelerare i percorsi necessari alle attività di bonifica generale, finalizzati, in particolare, alla rimozione e allo smaltimento di questo materiale, da realizzarsi da parte della società Syndial. In merito alle predette attività, si informa che, solo a seguito del definitivo completamento della caratterizzazione del CIC disposta dalla procura, si potrà procedere all'individuazione ed alla realizzazione degli interventi di bonifica più opportuni. A riguardo, è opportuno dire che nel corso di diversi incontri tenutisi con l'amministratore delegato della Syndial, nel sottolineare la criticità della situazione, sono state ribadite le prescrizioni già impartite in sede di Conferenza di servizi. In merito al CIC, la società ha dichiarato la più ampia disponibilità a collaborare con gli organi inquirenti al fine di accertare l'effettivo stato dei luoghi in cui il materiale è stato impiegato, nonché a farsi carico degli eventuali interventi di ripristino che dovessero rendersi necessari. Con riferimento, poi, alle implicazioni sulla salute pubblica, sono intervenuti anche il Ministero della salute e l'Istituto superiore di sanità, nonché il Dipartimento tutela della salute della Regione Calabria, con ARPA Calabria e rappresentanti degli enti locali, creando una vera e propria *task force*, volta ad approfondire le analisi ed indagini del caso. In base all'inchiesta della procura di Crotone, il conglomerato risulta essere presente in 23 aree, 4 delle quali interne al perimetro del SIN in questione. Per quanto concerne le altre, si fa presente che la Provincia di Crotone ha richiesto al Ministero dell'ambiente di procedere con decreto, ministeriale del 26 novembre 2002, all'estensione della perimetrazione del SIN, al fine di ricomprendere al suo interno tutte le aree oggetto dell'interramento delle scorie. Tale richiesta sarà posta all'esame della conferenza dei servizi di prossima convocazione. Per quanto concerne l'*iter* istruttorio relativo agli interventi di ripristino del sito, è giusto dire che Syndial fino ad oggi ha provveduto a presentare gli elaborati progettuali relativi alle aree ex Pertusola, ex Agricoltura ed ex Fosfotec, che hanno tenuto conto delle diverse prescrizioni impartite dal Ministero dell'ambiente al fine di assicurare la realizzazione di interventi maggiormente efficaci e cautelativi, nonché di definire il percorso più idoneo ad abbreviare i tempi della predisposizione e dell'esame degli elaborati richiesti. Riguardo poi alla salubrità delle acque nello specchio antistante la città di Crotone, si rappresenta che il Ministero dell'ambiente, in applicazione dei propri compiti istituzionali, scaturiti dalla legge n. 979 del 1982, conduce da quasi vent'anni un attento controllo sugli ambienti marini costieri italiani, attraverso programmi di monitoraggio svolti in collaborazione con le Regioni costiere. II penultimo di questi programmi, iniziato nel giugno 2001 e conclusosi nel gennaio 2007, ha previsto il controllo periodico e sistematico di acqua, sedimenti, molluschi, comunità plantoniche, comunità animali e vegetali dei fondali marini in 81 aree di indagine dislocate lungo tutte le coste italiane, tra le quali rientra anche l'area marina antistante il Comune di Crotone.

ha preso avvio il nuovo programma di monitoraggio, finalizzato in parte al proseguimento delle attività di controllo nelle suddette 81 aree di indagine, ma anche alla definizione di condizioni ambientali di riferimento e di livelli di contaminazione chimica recente e pregressa, alla estensione dei controlli ai popolamenti di macroalghe che popolano i fondali rocciosi, alla ricerca di nuove sostanze chimiche, come quelle incluse nella lista delle sostanze prioritarie e pericolose di cui alla decisione n. 2455/2001/CE, conseguente alla direttiva 2000/60/CE, nonché al controllo della diffusione di specie algali, anche bentoniche, produttrici di tossine. Ad ogni buon fine, si rappresenta che anche la bonifica delle acque prospicienti il sito industriale di Crotone rientra comunque nel programma di bonifica del SIN. Da ultimo, riguardo alla presenza della criminalità organizzata nel Crotonese, c'è da dire che questo è un dato abbastanza acquisito, anche processualmente. Va però aggiunto che l'attività investigativa per combatterla è stata notevolmente intensificata, molto più di quanto non sia avvenuto negli ultimi anni. A dimostrazione di ciò c'è proprio l'orientamento del Governo in tale direzione, che fa della lotta alla mafia una propria priorità, confermata dalle operazioni di polizia che sempre più frequentemente vengono portate a termine in questo territorio con ottimi risultati: e quindi la privazione della libertà personale, di soggetti dediti ad attività illecite e il sequestro di beni acquisiti con le stesse attività. Anche l'operazione denominata "Black mountains" è frutto di una di queste attività e, anche in questo caso, la magistratura, con 1'ausilio delle forze di polizia,

Signora Presidente, ringrazio il Sottosegretario anche se i contenuti della risposta all'interrogazione mi lasciano profondamente insoddisfatto. Di fatto

da un'azienda fondamentalmente controllata dalla mano pubblica, che per anni ha operato su quel territorio, nel quale non solo non si inizia

per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri si risponde all'interrogazione del senatore Vincenzo Maria Vita ed altri, n. 368, concernente manifestazioni di protesta ed episodi di occupazione di edifici scolastici in relazione alla legge n. 169 del 30 ottobre 2008, che ha convertito il decreto-legge 1°

in coerenza con l'imprescindibile esigenza di tenere in ordine i conti pubblici, tendono a restituire qualità, efficacia, efficienza e credibilità al sistema scolastico italiano, considerate le negative valutazioni della scuola italiana risultanti da indagini e studi condotti da autorevoli organismi nazionali ed internazionali. Di tale negativa situazione era d'altra parte consapevole anche la precedente gestione, come risulta dal Libro bianco sulla scuola dalla stessa pubblicato. Vanno inoltre tenuti presenti gli obiettivi posti dalla Strategia di Lisbona del 2000, al cui raggiungimento è necessario tendere. Alla luce del descritto contesto vanno quindi valutati i provvedimenti contenuti nella legge n. 169 del 2008 che, come rilevato dall'onorevole senatore interrogante, hanno suscitato reazioni sfociate, talora, anche in occupazioni delle sedi scolastiche. Fatta questa doverosa premessa, vengo alle domande poste dall'onorevole senatore interrogante precisando, innanzi tutto, che il Governo si è sempre mosso in una linea di ampia tutela del dissenso, purché lo stesso non assumesse forme contrarie alla missione educativa, che è a fondamento delle istituzioni scolastiche, e modalità contrarie alla normativa. Al fine di stemperare il rilevato contrasto tra il Governo e parti delle componenti scolastiche, il ministro Gelmini, per contribuire al miglioramento del confronto dialettico e del dialogo, già dal 4 dicembre scorso ha aperto un canale su "Youtube" confronto con i ragazzi attraverso videodomande o commenti che tutti possono inviare. Ogni settimana il Ministro risponde agli studenti sui temi della scuola, dell'università e della ricerca per spiegare le riforme senza filtri, in modo che ogni studente possa autonomamente farsi un'opinione sulle iniziative intraprese dal Ministero. In merito alla domanda diretta a conoscere se «denunce e identificazioni si configurino come repressive ed intimidatorie, in particolare nei confronti di ragazzi minorenni», il Ministero dell'interno ha comunicato quanto segue in relazione agli specifici episodi cui si fa riferimento nell'atto in discussione. Né a Padova né a Treviso sono state riscontrate occupazioni di edifici scolastici. Relativamente a Milano, il 3 novembre 2008, alle ore 7,55, il preside dell'Istituto magistrale "Agnesi" ha contattato telefonicamente il competente commissariato di pubblica sicurezza per segnalare la presenza, all'esterno dell'edificio scolastico, di diversi studenti muniti di megafoni. Peraltro, dopo circa 25 minuti, la centrale operativa del Comando provinciale dei carabinieri disponeva l'intervento di una pattuglia del proprio nucleo informativo presso lo stesso istituto, a seguito di una segnalazione di un assembramento di studenti che impediva l'accesso alla scuola. Le forze dell'ordine constatavano la presenza di alcuni giovani che incitavano gli studenti a protestare contro la riforma scolastica e si avvicinavano all'ingresso, ove un'insegnante era presente per agevolare l'ingresso di quegli studenti che intendevano entrare a scuola. Avendo la medesima insegnante respinto la richiesta dei manifestanti di mettere a disposizione un locale per tenere un'assemblea, a causa dell'indisponibilità del locale stesso (la palestra era infatti chiusa per lavori), gli stessi si portavano nel parco antistante l'edificio, dove venivano raggiunti da altri studenti provenienti dalla sede succursale. Lo stesso gruppo, intorno alle ore 8,50, dopo aver cercato di entrare nell'edificio (il portone era chiuso) riusciva ad entrare da un ingresso laterale (verosimilmente grazie all'aiuto di qualcuno presente all'interno). Nella circostanza veniva travolta un'insegnante, rimasta contusa ad un braccio. Successivamente, l'insegnante ferita ha sporto querela per lesioni personali. A Bologna la questura ha svolto un'opera di monitoraggio delle manifestazioni studentesche mantenendo stretti contatti con le autorità scolastiche che, peraltro, non hanno ravvisato la necessità di richiedere l'intervento delle forze dell'ordine, né hanno segnalato episodi di violenza o di danneggiamento. Peraltro, in occasione dell'occupazione della scuola elementare "XXI aprile" un deputato al Parlamento ha presentato un esposto-denuncia sull'eventuale sussistenza di illeciti penali in relazione al coinvolgimento dei bambini in occasione delle proteste. Il giudice per le indagini preliminari ha accolto la richiesta di archiviazione della procura. A seguito di ulteriore esposto-denuncia del medesimo deputato, l'autorità giudiziaria ha delegato la locale DIGOS a svolgere accertamenti circa le modalità con le quali sono state attivate le iniziative di protesta. A Roma, invece, il 27 e il 29 ottobre 2008 il dirigente scolastico del Liceo classico "Giulio Cesare" ha denunciato alla procura della Repubblica, nonché al commissariato di pubblica sicurezza ed alla competente competente stazione dei carabinieri, l'avvenuta e cessata occupazione dell'edificio scolastico da parte di studenti che hanno impedito agli insegnanti di svolgere l'attività didattica, segnalando che nel corso dell'occupazione gli studenti, oltre a non arrecare danni, hanno anche provveduto a tinteggiare gli ambienti occupati. L'autorità giudiziaria ha delegato le indagini ai carabinieri. Sempre a Roma, invece, nella prima mattina del 3 novembre 2008, una trentina di studenti ha occupato il Liceo "Dante Alighieri"; verso le 19 dello stesso giorno hanno desistito dall'occupazione ed hanno invece optato per una forma di autogestione. Nel corso degli eventi, che non hanno fatto registrare danni a persone o cose, il personale docente, gli impiegati e gli studenti dissociatisi dall'iniziativa hanno sostato all'esterno dell'edificio, così come i carabinieri dipendenti dalla stazione Prati, che non hanno proceduto ad alcuna identificazione.

risposta, ancorché assai tardiva. Non certo per sua responsabilità, Sottosegretario, tuttavia tardiva. tardiva. Il tempo, che è la variabile decisiva in quasi tutte le attività, anche in questo caso è tiranno: ha scavato, perché nel solco delle sue parole si rintraccia una risposta tempestiva forse qualche tempo fa, ma oggi un po' evasiva, anche alla luce di quanto avvenuto, da ultimo, proprio l'altro ieri, con

viene derubricato e vissuto come puramente repressivo da parte di migliaia di giovani che hanno un rapporto con la vita pubblica ancora incipiente e pieno di attese. Perché deludere queste attese?

Tante esperienze passate ce lo hanno insegnato: quando il rapporto con i movimenti (anche quando sono un po' estremi) un po' estremi) è finalizzato al dialogo e al confronto, persino dicendo dei no (non sto rappresentando qui un'astratta esigenza di dire sempre un accorato sì), allora il dialogo cresce e anche lo spirito riformistico di un Paese avanza. Quando invece un atteggiamento di tagli del sapere e delle spese per la cultura potrei fare un elenco infinito, ma non ve ne è bisogno - si aggiunge a un'ottica strettamente repressiva del movimento dei giovani, può emergere disaffezione, come infatti è successo, e le tante astensioni che crescono in Italia ad ogni tornata elettorale ne sono una dimostrazione. Astensioni e disaffezione verso la cosa pubblica che sono assai più gravi quando si è molto giovani di quanto non lo siano in età più adulta. è poi persino il rischio di violenze. La violenza, infatti, ci hanno insegnato illustri studiosi, si anima proprio così, cioè parte da qualche episodio, magari anche occasionale, e poi diventa una pratica che può costituire un pericolo effettivo. Ecco perché la sollecitazione degli interroganti all'epoca - e lo ribadisco qui, Sottosegretario - è di tenere conto che questo non è un problema finanziario: